*(PD)*. Signor Presidente, la 5a Commissione ha concluso questa notte i suoi lavori senza il mandato al relatore e quindi sono qui io a riferire dei lavori. ha concluso esprimendo un sentimento di rammarico, che devo dire ha unito tutti i Gruppi, ed anche il Governo, per non aver potuto effettuare una lettura compiuta del disegno di legge di bilancio.

Da parte delle opposizioni questo elemento è stato caricato comprensibilmente di aspetti anche di tipo polemico e critico nei confronti del Governo e della maggioranza, mentre da parte della maggioranza e del Governo si è obiettato che in un contesto di crisi di Governo, politicamente di fatto già aperta, sarebbe stato difficilmente comprensibile un dibattito di merito

Per quanto riguarda gli ordini del giorno è stato convenuto, sia da parte dei rappresentanti dei Gruppi che da parte del Governo, che non avrebbe avuto alcun senso impegnare su questo o su quel tema un Esecutivo che è già di fatto dimissionario.

che in qualche modo prendeva atto dell'impossibilità di procedere ad un esame e ad una votazione di tutti gli emendamenti. Si è convenuto, quindi, sull'impossibilità di concludere i nostri lavori con un mandato al relatore e d'altra parte i Gruppi di opposizione non hanno insistito sulla votazione, che sarebbe stata a quel punto un inutile esercizio, vuoi in ragione del calendario dei lavori d'Aula, vuoi in ragione del fatto che è stata già preannunciata la presentazione della questione di fiducia e che dunque gli emendamenti sarebbero comunque decaduti.

dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2611 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2611, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Vorrei spiegare due cosette in merito a quello che sta accadendo in Europa e anche in Italia, perché forse qualcuno ha perso il collegamento con il mondo esterno.

che la BCE stava comprando i titoli governativi tedeschi e non quelli italiani, quindi era normale che lo *spread* aumentasse.

- ciò avrebbe potuto indurre un aumento della instabilità sociale in altri Paesi europei che stanno già sperimentando forte resistenza al cambiamento alla vigilia di importanti elezioni del 2017. che il presidente emerito Giorgio Napolitano, che è stato il manovratore di questo Governo, venisse a riferire in Aula anche se non c'è il Governo e a rispondere se veramente in quei nove anni ha fatto gli interessi del Paese o quelli della massoneria.

Signor Presidente, finisce oggi la vita di un Governo che ha rappresentato un caso di scuola

infatti l'intervento svolto dal Presidente del Consiglio in quest'Aula per il suo insediamento, con le mani in tasca e rivolto alla tribuna ridicolizzando quest'Assemblea. Questo atteggiamento poi è proseguito nel corso della legislatura, imponendo al Parlamento una modifica per stravolgere la Costituzione che è stata approvata tra mille forzature, procedendo all'acquisto, mediante promesse mirabolanti, di numerosi parlamentari. Anche il provvedimento che stiamo discutendo oggi, il disegno di legge di bilancio 2017, procede nel suo *iter* senza alcuna discussione in Commissione, eppure siamo solo ai primi di dicembre e ci sarebbe stato tutto il tempo per apportare modifiche e correzioni, per discutere emendamenti che sarebbero assolutamente necessari per rendere il disegno di legge di bilancio il più corretto possibile; invece oggi siamo qui a votare anche questo provvedimento con la fiducia. Debbo dire che in dieci anni di attività parlamentare, anche come membro della Commissione bilancio, non ho mai visto una manovra finanziaria schifosa come quella che state per approvare.

perché vogliamo che si approvi questo disegno di legge di bilancio con l'augurio che si vada immediatamente a nuove elezioni per poterlo correggere tutto, perché è tutto sbagliato. Grazie ma ciò che vorrei fissare durante questo discorso è l'eredità pesantissima che ci lasciano le bugie e le chiacchiere del Governo Renzi. Si inizia con la legge di stabilità dell'anno scorso che ci lascia in eredità, per il 1° gennaio del 2017, tagli feroci a carico delle Regioni e della sanità: saranno 4 miliardi l'anno prossimo e 5 miliardi nel 2018 e nel 2019. Ma subentrerà sicuramente un Governo che, finalmente, anziché pensare alle *lobby* e alle banche (soprattutto alle banche, dove amministra il ministro delle riforme Boschi), penserà

di aiuti presi dalla fiscalità generale, ma soprattutto dal Sud. Noi non vogliamo un Governo del genere, non vogliamo un *Premier* che, ancora sotto scacco sconfitto, pubblica le ennesime *slide* dicendo che il debito pubblico è diminuito: dal 1871 a oggi abbiamo raggiunto il picco del rapporto debito-PIL,

quando in realtà non hanno fatto altro che incetta delle disponibilità liquide di tesoreria per fare un ennesimo annuncio. In realtà quello che ci lascia in eredità sono 100 miliardi di nuovo debito pubblico fatto solo per i *bonus*. Questo è stato un Governo estremamente tecnico. Abbiamo avuto un Ministro dell'economia e delle finanze che è stato voluto dal Fondo monetario internazionale e dalle banche. Abbiamo avuto un *Premier* che è stato finanziato, con il tramite per fare mance elettorali da una Commissione europea estremamente politica che voleva fermare il populismo e voleva fermare il popolo, ma non ce l'ha fatta. Ora se ne deve andare a casa immediatamente. È il popolo che lo ha chiesto, non è più solo il Movimento 5 Stelle. È stato veramente deludente vedere per l'ennesima volta le promesse sui bambini di Taranto tradite, le mancette date a De Luca non abrogate, perché almeno questo Governo poteva andare via con un minimo di decenza e con meno vergogna, con un po' più di pudore, ma non è riuscito nemmeno a fare questo. Non ha abbassato le tasse questo Governo, ma ha fatto solo dei favori alle banche: ha portato la deducibilità delle perdite su crediti da diciotto anni a un anno. Con questa maggioranza, prima con il Governo Letta e poi con il Governo Renzi, tutto il Partito Democratico è responsabile di questo fallimento: non solo Renzi, ma tutti i senatori e deputati del Partito Democratico che si sono piegati e hanno detto sì a tutti questi favori alle banche e alle grandi imprese, al saccheggio del Sud, al saccheggio delle imprese artigiane e delle piccole Tutto il Partito Democratico è responsabile di questo ennesimo tonfo. Noi abbiamo quindi responsabilmente presentato pochi emendamenti

2018. I risanamenti edilizi e tutti gli investimenti fatti sulle scuole, sulla ricerca, sullo sviluppo e per l'aiuto alle imprese erano previsti dal 2018 in poi, quando neanche più si potrà chiedere flessibilità. Hanno messo il nostro Paese all'angolo, ma per fortuna il popolo ha alzato la testa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Avremo un nuovo Governo e una nuova maggioranza e tutto questo verrà messo a posto. Basta fare una legge anticorruzione e smetterla di fare i favori agli amici degli amici; eliminare veramente gli sprechi

Ci dobbiamo liberare ed è il popolo che ha chiesto la liberazione da questo Governo, dicendo no a quella riforma costituzionale ed esprimendo così anche un voto politico.

di legge di bilancio in esame ha radici lontane e conclude una parabola che si è aperta in quest'Assemblea con un discorso dimenticabile, il primo fatto al Senato dal Presidente del Consiglio, che credo tutti ricordiamo: Grazie aveva in tasca anche un grande progetto che consisteva sostanzialmente nel radere al suolo

che accettavano un Presidente non eletto, ma - soprattutto - delle varie forze che, in buona fede e senza talvolta nemmeno chiedere uno strapuntino di Governo (parlo di tanti parlamentari come il sottoscritto), erano disponibili a fare una tregua per cambiare la situazione. Si sono battute altre strade. Quel discorso ci fece capire che sarebbe stato molto difficile inseguire quella prospettiva. aveva un sapore collodiano, in quanto ricordava un po' quei personaggi adolescenziali descritti da Collodi: Pinocchio redimibile, Lucignolo irredimibile.

la leva che ha azionato per cercare di prendere quel consenso, che nel Paese non c'era, è tutta contenuta nella manovra Questa è la manovra in cui si agita lo spettro dei favori a De Luca, è la manovra che mangia in una volta sola tutta la nostra residua flessibilità, ed è la manovra che a marzo dovremo ritoccare, perché ha problemi di coperture. Questa è la manovra che ha consentito a quotidiani amici di

e già alla prima trimestrale avremo la certezza di dover rimettere le mani su coperture tanto "bollinate", quanto inverificabili in questo momento e purtroppo verificabili da qui a tre mesi. C'è poi il secondo aspetto grottesco della manovra in esame. Alcune di queste promesse, quelle forse meno visibili sui titoli dei giornali,

con un'improntitudine - che ha una parentela con quelle mani in tasca del primo discorso fatto al Senato - la stessa notte, a mezzanotte, il Presidente del Consiglio, con la manovra finanziaria aperta, si dimentica - glielo deve poi ricordare il Capo dello Stato - che un Governo in carica, anche se il Presidente del Consiglio fosse Grimilde, la strega di Biancaneve innamorata della propria immagine allo specchio, dovrebbe chiudere la finanziaria prima di dimettersi. In un Paese normale è evidente a chiunque, ma non lo è al Presidente del Consiglio, che a mezzanotte si dimette con un discorso

che sarebbe ben paradossale che un Governo dimissionario - che peraltro tale non è, finché non si dimette davanti al Presidente della Repubblica - discutesse e perfezionasse la propria manovra di stabilità, dei pareri come se fosse un normale Governo; e la grande risposta che risolverebbe questa imbarazzante situazione è che un Governo dimissionario metta la fiducia: signor Presidente, un Governo dimissionario mette la fiducia! Questa è la logica che ci porta alla mattinata odierna. È chiaro che quando si hanno dei *leader* paradossali, colleghi della maggioranza, ad un paradosso bisogna giungere: era un paradosso rispondere emendamento per emendamento; è un paradosso ancora più grande chiedere la fiducia per dimettersi.

canto, non voglio dire che i mercati festeggiano la sconfitta del sì o le dimissioni del Presidente del Consiglio, perché sarei ingeneroso, ma ci sarà un motivo se la borsa, dopo aver in parte scontato l'idea che il no potesse vincere e che ci fosse una crisi di Governo, ha recuperato dai due ai quattro punti negli ultimi due giorni e se lo *spread* è sceso. Ciò sta a dimostrare che il giudizio dei mercati sull'attività di questo Governo non è quello che ci è stato raccontato per un paio di mesi prima di questa campagna referendaria.

e che il Senato ha un ruolo nella valutazione delle leggi e soprattutto della legge principale, che è ovviamente quella legata alla stabilità economica e finanziaria del Paese, il paradosso è che al Senato viene impedito di correggere tale legge, perché si deve correre a raccontare alla direzione del Partito Democratico che se l'Armageddon nei mercati e nelle borse non c'è stato, cercheremo di procurarcelo con un *auto da fè*,

Sono cose che fanno i sindaci dei Paesi piccoli, quelli che si convincono di essere diventati podestà perché in un momento di debolezza di quel Comune sono stati premiati da un voto elettorale. Il nostro caso, dal punto di vista psichiatrico, il fatto è più grave perché il Governo non è stato nemmeno premiato dal voto elettorale.

avrebbe mai pensato di riportarci in una tale condizione di rigidità di bilancio causata dalla diffusione dispersiva e a pioggia delle poche risorse di cui disponevamo per fare delle manovre più serie.

soprattutto il mio Gruppo che ha commesso l'imperdonabile errore di concedermi ben sette minuti per parlare. Io, invece, per andare incontro ai *desiderata* della

secondi. Dico questo con lieve ma non superficiale ironia, perché

e, naturalmente, dopo che si imponeva, come sempre nelle seconde letture, una discussione anche emendativa importante e seria per portare una manovra seria fino al termine.

E ben si poteva, tranquillamente, finire in quel modo. Ho ben presente il dibattito del Presidente della Commissione e di tutti senatori e del Governo, nell'Aula della Commissione bilancio, che mi conforta ancora, innanzitutto, sulla bontà della scelta popolare e poi sul *vulnus* istituzionale che, ancora una volta, è stato compiuto. Parafrasando, però, la prima frase del Presidente del Consiglio, dopo aver dopo aver compiuto il primo *vulnus* il primo giorno in cui si è presentato in quest'Aula, per fortuna per lui questo è l'ultimo *vulnus* che egli ha inferto all'istituzione Senato, volontà del popolo. Signor Presidente, il punto è davvero molto grave. Ci sono tutte le risorse all'interno di questa istituzione, dell'intero Parlamento, dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni, a tutti i senatori, perché esso venga sempre rispettato e si la coltre di bugie - bugie invece, pubbliche - sui modi e i termini dei lavori nelle aule del Parlamento, e del Senato in particolare. Io mi auguro che, a partire dalla prima legge del nuovo Governo, si torni a un modo ordinato, serio

si voleva dimostrare che il Senato è efficiente nel fare tutto in poche ore, dimostriamo anche questo. Dire che anche Usain Bolt, nei confronti dei tempi che ci sono stati assegnati,

bene. Signor Presidente, anche questo modo di tentare di condizionare l'attività del Parlamento non solo è inaccettabile sotto il profilo istituzionale, ma soprattutto non ha alcun riscontro. Lascino lavorare il Parlamento e poi le altre componenti della società, ivi compresi i mercati finanziari, valuteranno, sotto il loro profilo, quali sono le ricadute del nostro operare. Ma questo vale

per il 2017 l'indebitamento è di meno 2,3, che - sapete - poi è diventato meno 2,4, e cioè peggiore

signor Presidente, il debito pubblico, che è il vero problema che poi orienta tutto il contesto extraparlamentare,

i 100 miliardi di debito in più. Voglio ricordare a noi stessi che il debito è una grandezza di cassa e, dunque,

meno scalpitanti, meno urlate, più serene, più serie, più ponderate. In questo modo dare un contributo serio, per quanto riguarda la nostra parte, alla ripresa della nostra Italia, a un nuovo rapporto con le istituzioni europee europee e con i grandi problemi che in questo momento abbiamo, primo fra tutto quello degli istituti di credito, che va approcciato in maniera serena e

di legge di bilancio in esame è stato scritto meramente in funzione della campagna elettorale (è pieno di regalini), ma non siete riusciti a ingannare ormai più nessuno. I nostri cittadini hanno dimostrato di essere più saggi della loro classe dirigente e politica. E, infatti, hanno bocciato la vostra riforma che - secondo il Governo - avrebbe sanato tutti i mali del Paese. Vi è stato detto non serve assolutamente velocizzare il processo legislativo ma, semmai, alzare il livello qualitativo del mondo di fare le leggi e ciò che abbiamo avanti ne è il tipico esempio:

Questa sicuramente non è una buona legge. La sua finalità elettorale è fin troppo evidente e, per inciso, vi diciamo che

Sapete benissimo che per legge non si possono includere nel disegno di legge di bilancio interventi di natura settoriale o localistici e, invece, il testo è pieno di mance e mancette. È una manovra bellissima di clientelismo elettorale.

dice che puoi imbrogliare tanta gente per poco tempo oppure puoi imbrogliare poca gente per tanto tempo, ma non puoi imbrogliare tanta gente per tanto tempo. E qua - ahimè - Renzi ha fallito. Avesse letto un po' di vecchi adagi popolari,

Bene, quella parte meno istruita vi ha dato una *lectio magistralis*, cari professori: infatti, vi ha detto che non vuole una dirigenza politica così spocchiosa e arrogante e che deve tornarsene a casa. Tenete i piedi per terra.

Inoltre, i famosi meno istruiti vi hanno detto che non ne possono più di un Governo di bambinette e di bambinetti viziati. E vi ricordo che questa parte di popolazione si alza tutti i giorni per andare a lavorare. È quella parte di Paese che di questa questa manovra fatta in *deficit* pagherà almeno i due terzi dei costi. Sono gli italiani più poveri che non possono più pagare le cure sanitarie, che vanno spesso a mangiare alla Caritas

per fare posto a degli immigrati. Forse anche in questo caso Renzi ha capito poco delle dinamiche che vive una grande fascia di popolazione. Continua a raccontarci che il PIL cresce, ma noi vediamo che un italiano su quattro sta scivolando in fascia di povertà. Renzi continua a mettere soldi nelle politiche dell'accoglienza, al punto da chiedere in Europa maggiore flessibilità. Peccato che le politiche dell'integrazione abbiano miseramente fallito. La stessa Merkel, appena rieletta in questi giorni al congresso del suo partito, ha dovuto dire che non si può transigere sulla cultura locale. In Germania c'è la legge tedesca e non la Sharia e le politiche dell'accoglienza devono rispettare senza regole, le leggi tedesche. L'ha capito anche la Merkel. Non l'hanno capito il Governo e il suo Grazie Renzi si sarebbe dovuto chiedere perché gli italiani continuano a non fare figli, nonostante continui a dire che eroga *bonus* a mamme e *bebé*, continuano a essere più precari, più poveri della generazione precedente e, addirittura, ad abbandonare affetti e nipoti per vivere all'estero, perché con le pensioni da fame in Italia non ce la fanno più.

Grazie ci fanno credere che siamo noi a scegliere, ma in realtà ogni riga di codesto atto non è altro che il risultato dell'asservimento dello Stato ai vincoli di bilancio europei, che ci hanno totalmente privato della nostra sovranità in favore dei mercati. D'altronde è il nostro stesso Governo che, nella relazione al disegno di legge costituzionale, confessa che negli ultimi anni forze non meglio precisate hanno imposto la trasformazione della nostra stessa forma di Stato e di conseguenza ormai tutto il resto deve essere improntato a questa illecita trasformazione. Per citare la frase per intero: «C'è l'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alla recente evoluzione della *governance* economica europea e alle relative e stringenti regole di bilancio». Pensate che è lo stesso Governo a definirle stringenti. E queste regole stringenti a chi sarebbero utili? Di certo non al popolo italiano, considerando che nel disegno di legge di bilancio per la lotta alla povertà sono stati stanziati soltanto 500 milioni e che a partire dal 2019 scenderanno a 300; considerando che un minore su tre è a rischio povertà e di esclusione sociale; considerando che nel nostro Paese la percentuale di giovani che abbandonano gli studi fermandosi alla licenza media supera la media europea. Persino gli investimenti pubblici per i prossimi tre anni sono ai livelli più bassi di sempre (pari al 2,2 per cento del PIL) ed è chiaro, invece, che è proprio questo tipo di investimenti ad agire come moltiplicatore della crescita economica. Non potete neanche più trincerarvi dietro lo *slogan* che le tasse sono diminuite, perché lo stesso ISTAT ha affermato che la pressione fiscale è aumentata aumenterà pure nel 2017, e ci si troverà di fronte un probabile aumento dell'IVA oltre il 26 per cento un Governo che si vanta tanto di voler dare un forte peso alle autonomie locali e poi viene fuori che, a ben vedere, le Regioni avranno 600 milioni in meno per provvedere al loro comparto sanità. Solo qualche briciola di elemosina si trova qua e là, mentre una voce di spesa non scompare mai ed è il finanziamento statale alle scuole private. Al contrario, vengono previsti *bonus* *una tantum*, i classici finanziamenti a pioggia, senza avere una vasta visione d'insieme e investire, invece, in un sistema di servizi socio-educativi che possano davvero fare la differenza. È una manovra che vale 27 miliardi di euro di cui oltre 10 miliardi sono in *deficit*. Quindi, se il popolo ne esce sofferente, povero, gravato da tagli alla scuola e alla sanità, e se gli investimenti pubblici non riescono a decollare con tanto di conseguenze nefaste sull'economia, a chi esattamente gioverebbero le "politiche stringenti"? Da qui mi viene il dubbio che i grandi protagonisti siano solo i grandi mercati finanziari, perché le politiche neoliberiste europee debbono avere sempre la meglio; politiche che hanno impoverito la nostra società, depresso l'economia e non hanno affatto risolto il problema del debito pubblico, che è addirittura aumentato. Ormai non solo siamo depauperati del potere di manovra, ma addirittura non si potrà neanche più discutere effettivamente di questa manovra a causa di una fantomatica fiducia tecnica, con il solo risultato che non ci sarà spazio per le modifiche e i senatori non si potranno rendere portavoce delle istanze del popolo, che è ciò su cui si fonda il nostro mandato. Il Parlamento viene espropriato delle proprie funzioni a colpi di fiducia, tanto per cambiare. Tutto ciò che era rimasto irrisolto alla Camera tale resterà e tutte le belle promesse fatte dal *Premier* che avrebbero dovuto confluire nel suddetto resteranno quello che sono sempre state fin dall'inizio: propaganda, una propaganda che è sempre stata basata su dati di crescita irrealistici, resa ancora più nefasta dalla cancellazione delle clausole di salvaguardia. Nessun cenno si rileva alla pesante deindustrializzazione che ha prodotto negli ultimi anni un elevato numero di disoccupati, facendo precipitare sempre più verso il baratro lo strategico settore manifatturiero. Anzi, la crisi imperante è servita come alibi per smantellare i diritti dei lavoratori, mentre quello che il popolo chiede davvero è che ci possano essere

c'è un'area di crisi industriale che conta un bel pezzo della produzione nostrana che scientificamente viene dismessa nel silenzio delle istituzioni. Non ci sono che briciole per il Sud, fatta eccezione per qualche mancetta qua e là, nessuna politica espansiva. Al contrario, si ha un'ulteriore spinta alla precarizzazione del mercato e del lavoro, ma nessuna crescita e nessuna riforma del sistema pensionistico. in ultimo, non posso che parlare di quello che è il MES; è certo che, se non avessimo contribuito con un esborso di 125 miliardi di euro per la quota che l'Italia deve corrispondere per l'istituzione del MES, mantenendo il nostro potere sovrano di autogestione, molte carenze avrebbero potuto essere sanate. E non sono solo quei 125 miliardi a pesare, quanto il fatto che, senza

Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di bilancio di cui oggi ci stiamo occupando ha iniziato il suo *iter* alla Camera, dove è stato approvato con l'apposizione della fiducia da parte del Governo, con la chiara convinzione che qui in Senato si sarebbe provveduto a dare il giusto completamento a un testo che, in tutta evidenza, risulta essere lacunoso e certamente non all'altezza di potersi definire una buona legge di bilancio. L'esito del *referendum* del 4 dicembre ha adesso generato una tale spropositata fibrillazione che anche in Senato il Governo si accinge a porre la fiducia, vanificando qualunque tentativo di miglioramento del testo. Ora, pur rendendoci responsabilmente conto della necessità del momento (che è quella di scongiurare l'eventualità dell'esercizio provvisorio) e anche alla luce delle annunciate dimissioni del Presidente del Consiglio, Consiglio, non possiamo esimerci dal dire che meglio si sarebbe fatto a evitare la fiducia tecnica e bene si sarebbe fatto, invece, a dare qualche giorno di tempo in più a quest'Assemblea per consentirle di apportare le necessarie modifiche che avrebbero reso il testo più accettabile e in grado di venire maggiormente incontro alle esigenze e alle tante aspettative dei cittadini. Ci sembra che il ricorso alla fiducia tecnica non sia un buon metodo di lavoro, soprattutto quando costituisce un epilogo per nulla calcolato. Non era questo che si attendevano i deputati alla Camera quando hanno deciso di votare la fiducia sul primo passaggio. Essi infatti sapevano, credevano e confidavano sul fatto che in Senato il testo sarebbe stato migliorato. Quindi, signor Presidente, come già ieri è stato detto più volte in quest'Aula, ritrovarci qui con un testo lacunoso, con una ingiustificata fretta, con il rischio di varare una legge di bilancio che potenzialmente potrebbe contenere anche degli errori non è certamente quello che desideravamo. Non vi è alcun dubbio che i mutamenti costituzionali informali, prodotti allo scopo di arginare fenomeni di ostruzionismo, comportano il venir meno del requisito della condivisione, che - a nostro modo di vedere - è un valore e non un «fastidio». Ebbene, con l'apposizione della fiducia tecnica mi sembra si voglia non solamente imprimere una non necessaria accelerazione ai lavori parlamentari, ma anche evitare espressamente, ancora una volta, la condivisione dei contenuti di questo disegno di legge di bilancio. Peraltro, si badi come il voto del 4 dicembre abbia manifestato la disapprovazione che il popolo nutre nei confronti della compressione della rappresentanza parlamentare. Il Senato eletto dal popolo è stato considerato un valore. è stata presentata come un'operazione di riduzione dei costi della politica: è stata letta, invece, dal popolo come una riduzione degli spazi di democrazia. Ora, se al Parlamento si continua a sottrarre la funzione legislativa con lo spostamento della centralità della formazione delle leggi dal Parlamento al Governo (in questo caso, con il maxi-emendamento dell'Esecutivo), non si va nella direzione indicata dai cittadini, della cui volontà dobbiamo essere rispettosi. Cari colleghi, qui siamo di fronte a una condizione anomala che, progressivamente, ha invaso la vita parlamentare, con la complicità di tutti quelli che hanno esasperato il concetto di «governabilità», a tutto discapito del ruolo del Parlamento e della democrazia. Certamente il mutamento radicale della politica italiana degli ultimi vent'anni non può che riverberarsi sulla democrazia parlamentare. Tuttavia, accompagnare tale cambiamento da parte del Parlamento senza consolidare funzioni nuove che bilancino quelle costrette a una compressione, come nel caso delle funzioni di indirizzo e controllo, significa condannare la funzione parlamentare, direttamente connessa con il sentimento e la qualità della democrazia di una Nazione, a un declino senza ritorno. Ecco perché avremmo voluto che questa legge di bilancio fosse stata trattata diversamente. Ecco perché avremmo voluto che le prerogative parlamentari non fossero state compresse una volta di più. si pensa? Si pensa che questo Senato sia così carente di responsabilità, al punto da far rischiare al nostro Paese l'esercizio provvisorio? Sono certo che non sarebbe accaduto. Con qualche giorno in più e lavorando sodo, credo che la Commissione bilancio avrebbe potuto licenziare un testo migliore e più condiviso ma, soprattutto, un testo con cui rispondere alle emergenze, la cui soluzione era stata promessa già a Montecitorio. È il caso - per esempio - dei precari siciliani che dal 1° gennaio, in assenza di proroga, andranno a casa, mettendo in seria difficoltà anche l'operatività di tanti enti pubblici. Eppure era stato promesso che, con il passaggio della legge di bilancio in Senato, il problema sarebbe stato risolto. Come si pensa di affrontare adesso il dramma di 22.000 famiglie? Purtroppo dovremo accontentarci del frutto zoppo di una fiducia tecnica. Peccato! È un'occasione sprecata anche per dare una risposta adeguata al segnale eloquente che il popolo ci ha trasmesso domenica. La gente ha desiderio di democrazia, ha desiderio di partecipazione e la vuole esercitare attraverso i propri rappresentanti, per i quali chiede spazi, agibilità, libertà di movimento e possibilità di trasferire le proprie istanze in ambito parlamentare:

Lega Nord non ha mai votato la fiducia a questo Governo e naturalmente non lo farà nemmeno in questa occasione. È paradossale affrontare quest'oggi una discussione sulla fiducia a sostegno a un Governo dimissionario, che è stato sfiduciato e bocciato dagli italiani. Vorrei chiarire che la responsabilità della attuale situazione di incertezza è di un'unica persona: l'attuale presidente del Consiglio dimissionario Matteo Renzi. È stato lui che, nel 2014, ha voluto cambiare il Presidente del Consiglio, prendendone il posto. È stato lui che ha voluto varare una riforma costituzionale a senso unico, imponendo attraverso il Governo al Parlamento una legge che divideva al Paese. È stato lui che ha creato un caos a livello di leggi elettorali, impedendo di fatto una situazione chiara, in vista delle prossime elezioni. È stato lui che ha deciso di tenere il *referendum* in piena sessione di bilancio. Sia chiaro, quindi, a tutti gli italiani che, se ci troviamo in questa situazione di emergenza, non è

che lo ha sempre assecondato nei suoi deliri di onnipotenza e nelle sue manie di grandezza. E come ha governato Renzi? Ha governato pensando di poter comprare il consenso, di poterlo comprare con i *bonus*, con le mance, con il voto di scambio alla De Luca, con l'arroganza. Ma i cittadini hanno bocciato questo metodo di governo. E, di fronte alla sua proposta di semplificare la democrazia con il suo impegno di ridurre i i cosiddetti costi della politica e in cambio ottenere dai cittadini un mandato pieno senza permettere più loro di eleggere i propri rappresentanti, il popolo ha risposto di ha risposto di no. Non vuole farsi comprare da Renzi, perché il proprio diritto di voto non è in vendita e lo ha manifestato nella consultazione referendaria. Cosa ci lascia Renzi alla fine di questa lunga esperienza di mille giorni? 106 miliardi di debito pubblico in più, perché il tentativo di comprare il consenso degli italiani ha rappresentato un costo per tutti noi e per le future generazioni. generazioni. Il Presidente del Consiglio lascia un Paese in ginocchio, al di là della propaganda con la quale ha tentato di oscurare la realtà nei mille giorni: una situazione migratoria fuori controllo - e credo che nessuno possa negarlo - un sistema bancario al collasso, con rischi immediati gravissimi; una disoccupazione alle stelle; tanta, troppa sofferenza nelle famiglie italiane. Questo è ciò che lascia Matteo Renzi nel Paese: giovani arrabbiati senza fiducia nel futuro, pensionati che hanno paura di perdere i propri risparmi e le proprie certezze. Questa è l'eredità del Governo Renzi:

basta Renzi! E diciamo finalmente anche noi per l'ultima volta: basta Renzi! si chiuda questo capitolo di cinque anni in cui i Governi si sono avvicendati attraverso giochi di palazzo; la parola passi ora al popolo al più presto; i cittadini tornino a essere protagonisti della nostra democrazia con l'unico modo democratico e legittimato, che può far sì che il prossimo Governo li rappresenti realmente, e cioè attraverso il voto. Basta Renzi! Subito al voto. *(Applausi Signor Presidente, il concetto di fiducia tecnica è un po' strano e dà l'idea del tentativo di rivestire in qualche modo qualcosa che non sta nelle regole, perché è fuori dal mondo che un Governo dimissionario chieda la fiducia

che andasse a sbattere, perché non ha voluto tenere conto delle tante voci che in questi anni chiedevano una diversa gestione dei problemi: voci interne al suo stesso partito e voci diffuse nel Paese. questo epilogo è un po' grottesco: un Governo dimissionario che chiede la fiducia per superare indenne la prova dell'Aula

un di più di modestia, una maggiore umiltà nel trattare problemi enormi che sicuramente non sono tutti nati da poco, ma che tutti abbisognano di cura

negato. Guardando a come ci si sta muovendo in questi giorni,

persone che ho conosciuto, abbandonate nelle mani della criminalità organizzata da parte di un Stato che li invitava a denunciare; mi riferisco a persone che si ritrovano a quarant'anni non solo senza un lavoro, ma senza una credibile prospettiva di trovarne Mi riferisco a malati cui sono negate le cure; mi riferisco a malati cui è negata la diagnosi; mi riferisco a donne gravide cui è negata la possibilità di partorire vicino casa, trasferendo

ed è stato sostenuto dallo stesso, anche perché, se non lo avesse sostenuto, il presidente Crocetta non avrebbe resistito più di un paio di giorni nelle condizioni in cui si trova, visto che è sospeso a un filo. Al di là di questo, il problema non è solo siciliano. Ho avuto contatti con miei connazionali di diverse Regioni e vi assicuro che questa maggioranza non è ben vista sul territorio, ovviamente laddove fosse necessario sottolinearlo, visti i risultati del *referendum*, che è stato politico. Attenzione: moltissimi italiani hanno rigettato il tentativo di accentrare troppo potere sul Governo e quindi hanno espresso un voto consapevole dal punto di vista tecnico. Ma molti italiani hanno comprensibilmente detto no a un Governo che - come accennavo all'inizio - guidava il Paese come se si trattasse di un motocicletta,

Ma a quegli italiani di cui parlavo prima, quelli senza lavoro, quelli senza cure, quelli che pensano di andare in pensione dopo quarantaquattro agli edili, che andranno in pensione quando non saranno già più in condizione di tenere in mano gli attrezzi del mestiere, chi ci pensa? Non Renzi e, temo, non una buona parte del Partito Democratico (francamente, penso che alcuni ci penseranno). Il Governo non doveva chiedere la fiducia; dovevamo andare responsabilmente all'esame di questo disegno di legge, affrontando quello che l'ordinamento prevede, anche l'esercizio provvisorio, perché no? È previsto: non un Governo tecnico, un esercizio provvisorio. È previsto dall'ordinamento.

per tentare di riparare ai danni causati dalla buona scuola: fondi stanziati per il potenziamento dell'organico dell'autonomia,

dovrà attendere, come dovrà attendere l'intera categoria dei docenti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale. Infatti, nonostante le forze di maggioranza abbiano sbandierato la volontà di sanare lo stato di precarietà di questo corpo docente,

rispettivo stanziamento di fondi, mentre alla ricerca rimangono gli spiccioli. È infatti chiaro, ormai, che l'intento di questo Governo fosse quello di introdurre in Italia il modello americano

tutto è nelle mani di una fondazione futura, non si sa come saranno reclutati i ricercatori e non si sa se il progetto resterà di utilità pubblica o se, gradualmente, finirà nelle mani e tra le fauci delle multinazionali del farmaco. Nulla si sa di come saranno gestiti i dati gestiti i dati genetici - i cosiddetti dati genomici - che sono un *big affair*, oltre che un *big data* da gestire.

il diritto di utilizzare i ricavi della bigliettazione e sottraendo queste risorse, preziose per la tutela e la valorizzazione non solo del Colosseo e dell'area di Pompei ma anche dell'area archeologica centrale di Roma, del Palatino e di tutte le aree circostanti.

di questi siti, ai quali giustamente era stata riconosciuta per gestire autonomamente e con risorse proprie la tutela e la valorizzazione di queste aree archeologiche e di questi siti culturali importantissimi. Si tratta di uno scippo bello e buono da parte del Ministero.

È quindi legittimo pensare che questa norma *ad hoc*, che sottrarrà Ales ai vincoli di contenimento della spesa, non farà altro che dare linfa ad una procedura

tutelare e valorizzare il nostro patrimonio artistico. Questa è la legge di bilancio che ci lascia in eredità il Governo Renzi, fatta non solo di "marchette", ma anche di "scippi" ai danni della scuola, dell'università e della nostra amata cultura. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, la fine del Governo Renzi è l'occasione per tirare le somme, non solo di questo disegno di legge di bilancio, ma della politica economica di questi mille giorni del suo Esecutivo. Le valutazioni sul triennio precedente si possono fare serenamente, perché siamo in possesso dei dati assestati, mentre le valutazioni sul triennio previsionale 2017-2019 sono soggette alla inaffidabilità a cui ci hanno abituato le precedenti stime di questo Governo.

Invece, il voto è slittato sino all'inizio di dicembre e questa è un'ulteriore prova di come, ancora una volta, si volessero utilizzare le misure economiche per creare facile consenso. Così non è stato. Il Paese ha dimostrato di non avere bisogno di mance, di *bonus* o di altre misure *una tantum*. necessita, al contrario, di condizioni che creino certezze e fiducia, in chi risparmia, in chi investe e in chi consuma: tutti gli indicatori di questi comportamenti sono ai minimi storici. L'Italia ha avuto la fortuna di beneficiare delle politiche monetarie espansive della BCE e di un *quantitative easing* in grado di regalare, in tre anni, al nostro bilancio più di 24 miliardi di euro di minori oneri sul debito pubblico. Grazie all'azione della Banca centrale di Francoforte si sono avuti inoltre riflessi positivi sia sul PIL, sia sull'avanzo primario. In assenza di questi interventi, il rapporto tra debito e PIL sarebbe ora al 145

100 miliardi di euro in più rispetto al febbraio 2014, 305 in più rispetto al Governo Berlusconi. Siffatti numeri abbiamo voluto ribadirli perché, come già sottolineato in altre occasioni, questo autentico regalo della Banca centrale sta per finire. I dati sull'inflazione in rialzo nel resto d'Europa non consentiranno al governatore Draghi ulteriori politiche espansive oltre la metà del prossimo anno. Qualsiasi Governo vada ad insediarsi il prossimo anno, dovrà quindi affrontare una manovra correttiva dei conti pubblici, probabilmente già dalla prossima primavera. Così come il calo di fiducia nel nostro Paese è testimoniato dai dati sulla bilancia dei pagamenti dell'ultimo anno forniti dalla Banca d'Italia: tra il settembre 2015 e il settembre 2016 si è registrata una fuga di capitali italiani verso l'estero per 82,4 miliardi; al contempo si è registrata una diminuzione degli investimenti esteri in Italia per 86,6 miliardi. Il risultato è che 169 miliardi sono fuggiti dall'Italia. Quindi, i mercati hanno dimostrato di non avere alcuna fiducia nelle scelte economiche del Governo Renzi, scelte fatte di *una tantum*, di *deficit* in entrata e di *bonus* in uscita. *Una tantum* si registrano anche in questa manovra, con quasi 6,5 miliardi di condono fiscale e circa 2 miliardi di anticipo - di dodici anni - dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione, con un *deficit* di 12 miliardi, per fare più spesa per l'accoglienza migranti, che è stato l'unico e vero motivo del contendere con la Commissione europea e con un vasto elenco di piccoli interventi localistici o microsettoriali che evito di citare tanto è lungo. Ripercorrendo le politiche economiche renziane, il peccato originale è stato proprio il *bonus* di 80 euro, una elargizione completamente iniqua dal punto di vista fiscale e sociale, fatta per fidelizzare una precisa fascia di elettori a ridosso del voto delle elezioni europee. Si sono accontentati quasi 10 milioni di contribuenti, dimenticandosi degli altri 30 milioni, ma si è commesso un atto di ingiustizia, perché, prima, bisogna dare qualcosa a chi ha meno, poi, eventualmente, dare a chi un reddito lo ha già. Voglio ricordare che il trattamento pensionistico minimo è fermo a 501 euro al mese, cioè ancora il vecchio milione di lire a cui lo aveva portato il presidente Berlusconi. L'Italia ha bisogno di uno *shock* fiscale, di una riduzione delle imposte importante, che al contempo allarghi la base imponibile, accompagnata da una energica riduzione del costo dello Stato. In realtà, in questi tre anni, la diminuzione della spesa pubblica è stata sopportata soprattutto dagli enti territoriali e dai servizi resi sul territorio. Lo Stato centrale non ha sostanzialmente diminuito il proprio peso, così come non è diminuito il peso della struttura e dei vincoli della pubblica amministrazione, principale freno alla crescita del Paese. Il saldo di questi tre anni vede, per effetto delle manovre di Renzi, una crescita della spesa per 42 miliardi di euro e un aumento delle tasse per 5 miliardi. In particolare, si è aumentata la spesa corrente, che nel 2017 vale il 93 per cento della spesa complessiva, al netto della spesa per interessi. Il prossimo anno, in conseguenza della manovra, si raggiunge la cifra *record* di 861 miliardi, cioè 40 miliardi in più rispetto al dato assestato del bilancio 2016, certamente, risultato del peso complessivo dell'onere del debito pubblico, ma anche conseguenza dell'aumento di spesa. Le spese finali aumentano di 9,4 miliardi rispetto al bilancio a legislazione vigente. Al di là dei proclami, quindi, la diminuzione delle tasse non c'è stata. I dati che ogni volta ci venivano presentati riguardavano un mancato aumento delle tasse, di volta in volta fortunatamente scongiurato. Nelle previsioni del bilancio in esame le entrate aumentano di 2 miliardi rispetto al bilancio previsionale a legislazione vigente e di quasi 6 rispetto a quello assestato del 2016 e questo nonostante la disattivazione della clausola di salvaguardia sull'IVA che vale poco più di 15 miliardi.

dicendo che pertanto si può parlare al massimo di un mancato aumento di tasse, peraltro previste dallo stesso Governo; mancato, per ora. Questi sono numeri, scritti nero su bianco, che preoccupano. Gli italiani, ormai sanno distinguere le bugie dalla verità, il racconto renziano di un'Italia idilliaca e il risveglio nella difficile realtà L'eredità che lascia al Paese questo Governo è pesante, perché ha mancato di mettere in sicurezza i conti pubblici, sfruttando le contingenti politiche monetarie favorevoli, perché non ha investito su un Paese che chiedeva di crescere e diventare più moderno. Chiunque vada al Governo avrà quindi un compito arduo, più arduo di quanto fosse nel 2014, quando è iniziata la disastrosa avventura di un Esecutivo non eletto di cui gli italiani non sentiranno la mancanza.

Dai banchi vuoti della maggioranza assistiamo a un silenzio assordante. E dire che la maggioranza ha la responsabilità di avere fornito questo strumento di programmazione finanziaria per il Paese. Nessuno ha trovato forza, coraggio, volontà per potere esprimere

dello stato in cui versa il Paese e di ciò che si intende fare per superare i punti di criticità: il PIL allo 0,8 per cento anziché al'1,1 così come era stato programmato, gli effetti che ha prodotto e come si intende dare dare risposta ai bisogni che, durante l'anno trascorso, si sono appalesati, come si intende fare uscire il Paese dalla sacca di crisi, di recessione e di larga disoccupazione. Questa è l'esemplificazione piena di quello che è stato il renzismo in Italia in questi anni: tanta propaganda, tanti proclami, nessuna sostanza. Ciò che è avvenuto domenica scorsa nelle urne, con una larghissima partecipazione popolare a un *referendum* che era di natura costituzionale e che ancora ci si attarda a leggere semplicemente come la risposta a un quesito di tipo costituzionale, è invece il segno vero, forte e determinato di quanto fallimentare sia stata la politica economica e dell'occupazione di questo Governo. Come si fa a non leggere i dati della scorsa domenica come il grido di dolore delle fasce più deboli della nostra popolazione? Come si fa a non comprendere? Sento ancora analisti dire che c'è una parte del Paese che non ha capito il progresso, che si sono scontrate le forze della conservazione contro le forze del progressismo e del guardare avanti.

che non ne possono più di un'attività di Governo che guardi agli interessi finanziari forti, un Governo che parla di buona scuola e realizza la peggiore scuola mai avuta in Italia, che parla di attenzione ai giovani e pensa di conquistarli con le mance anziché programmare il loro futuro con un piano di occupazione e di risveglio. Non vedete che, partendo dal Trentino fino ad arrivare a Portopalo, le percentuali del vostro "sì" andavano assottigliandosi man mano che si appalesavano i fallimenti delle vostre politiche? Fino ad arrivare a quell'Agrigento del Ministro dell'interno, che, nonostante il sì fosse appoggiato da Ministri, da Presidenti di Commissioni parlamentari e dai sindaci delle città, per cento, quasi a dire: ma chi se ne frega delle vostre architetture costituzionali che debbono servire per aumentare il potere di Renzi, del *Premier*, o per riorganizzare i vostri assetti interni di potere!

Questi sono i problemi. E questa legge di bilancio, ancora una volta, nel solco della continuità delle vostre politiche degli ultimi tre anni, non affronta nessuna di queste problematiche. C'è una cosa di cui sono contento, signor Presidente, e credo che anche lei, per appartenenza e per sentimenti meridionali, ne potrà essere contento: da domenica in poi, nessuna forza politica potrà far finta di non comprendere il malessere e la necessità di una forte ripresa di politiche a sostegno dello sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Lo sappiano tutte le forze politiche che siedono in quest'Assemblea: prescindendo dalla reale esigenza politica dei territori, si perde (e voi avete clamorosamente perso), ma perderanno in futuro tutti coloro che faranno finta di non vedere la sofferenza del popolo italiano, che faranno finta di non vedere un'Italia che ancora cammina a doppia velocità, faranno finta di non vedere o pensino di poter risolvere il problema imbonendo le popolazioni, facendo i comizi elettorali, dicendo che faranno i ponti sugli stretti o o prospettando un roseo futuro basato soltanto sulle buone intenzioni. No, non sarà più lastricata di buone intenzioni la strada che porterà al successo elettorale e quindi alla conquista del governo di questo nostro Paese: è arrivato il tempo della serietà, il tempo dell'assunzione di responsabilità piena. Non è possibile, ancora una volta, in questi giorni, assistere a questo doppio binario. Saluto la serietà istituzionale, l'atteggiamento forte che ci tutela, anche sul piano della finanza (basti vedere l'andamento delle borse), l'assunzione di responsabilità del nostro Presidente della Repubblica. Eppure, a fronte di un atteggiamento che ci consente di attraversare questo momento molto delicato con le istituzioni europee, con le istituzioni mondiali, con gli operatori finanziari, nella tranquillità di sapere che l'Italia, in ogni caso, ha una guida autorevole e seria,

senza legge elettorale. Per inseguire che cosa? Il facile consenso. No signori, no amici miei, no cari colleghi, non è più tempo del facile consenso e del populismo a basso costo: è il momento dell'assunzione di responsabilità. Il nostro Paese, la nostra Italia oggi ha bisogno che ognuno di noi svolga il proprio piccolo, grande ruolo per superare questi momenti di grandissima difficoltà e fare in modo che la nostra presenza nel contesto internazionale, ma soprattutto in riferimento ai bisogni del nostro Paese, possa dare una risposta responsabile, forte e seria. Tornando nei nostri collegi e nelle nostre case, come possiamo non dare il segno di avere capito? Come possiamo non dire ai nostri cittadini, ai nostri italiani, che

Gli italiani sono tornati a votare, quindi non è vero che c'era una disaffezione per il voto. C'era la disaffezione rispetto a una politica

potuto comprendere che il loro sì o il loro no determinava intanto un effetto immediato, quello di salvaguardare un sistema democratico e la propria sovranità popolare, si sono recati in massa a votare per determinare ciò che hanno ritenuto essere meglio per il proprio futuro democratico. Alla stessa maniera, il modo di impostare le politiche e di affrontare i problemi dovrà essere, dal punto di vista della realtà, concreto e determinato. non se ne può più. Nella quotidianità dei rapporti si è strozzati da un sistema bancario che impedisce l'accesso al credito e, se malauguratamente il rapporto con il credito genera contenzioso, porta all'esasperazione e addirittura a gesti di autolesionismo perché non si riesce a dialogare con il sistema bancario con il sistema bancario e con un sistema istituzionale sempre lontano. Le riforme proclamate non hanno determinato vicinanza tra i cittadini e le istituzioni. Per questo, signor Presidente, siamo decisamente contrari a questo disegno di legge, nel quale non abbiamo potuto inserire gli elementi che riteniamo fondamentali e rinviamo questo nostro impegno ai futuri momenti, che ci auguriamo possano

chi non riesce a dare il segno concreto della costruzione del futuro è contro non solo i nostri giovani ma anche contro il nostro Paese. Per questo voteremo no alla fiducia a questo Governo. il nostro è un no sul merito e sul metodo che avete utilizzato per portare in quest'Aula il disegno di legge di bilancio. Il metodo lo conosciamo tutti e ne abbiamo parlato ieri. Avete totalmente sbagliato per l'ennesima volta: avete sbagliato il metodo e il modo di approcciarvi al Senato della Repubblica.

coperto di cenere, avrebbe dovuto cercare di iniziare un rapporto tra istituzioni della Repubblica italiana. Il problema è che, ancora una volta, si è voluta utilizzare l'arroganza,

ascoltare la fiducia che darete a questo Governo. Si poteva fare quello che avevamo detto:

non per il bene del Senato, non per Renzi che ha dato le dimissioni (e chi se ne frega delle sue dimissioni), ma per il bene degli italiani, per il bene di tutte quelle persone che si aspettavano e si aspettano qualcosa da questo disegno di legge di bilancio per tutte le promesse che avete fatto in campagna elettorale. Infatti, in campagna elettorale, per portare a casa i milioni di voti che avete ottenuto (perdendo), ne avete fatte di promesse:

sappiamo benissimo che buona parte di quelle promesse, purtroppo, dovevano passare dal Senato. Le modifiche dovevano passare in questa Assemblea. E quindi, mettendo la fiducia, avete disatteso le aspettative degli italiani, di 28 milioni di italiani a rischio di povertà, di categorie intere di precari che in questo momento stanno aspettando e ci stanno ascoltando. Alcuni, anche questa notte, ci dicevano: «Cambiate qualche cosa». Non possiamo cambiare niente, cari amici, perché loro hanno messo la fiducia. Non possiamo cambiare niente, cari italiani, perché loro hanno messo la fiducia e non vogliono cambiare niente!

di pezza. Questo lo dobbiamo dire agli italiani. Diciamolo agli insegnanti precari, ai precari dei Vigili del fuoco, alle Forze dell'ordine, ai dipendenti della pubblica amministrazione. Diciamolo a tutte quelle persone che in questo momento stanno ascoltando e aspettano qualcosa. Diciamolo agli agricoltori, diciamolo anche alla Coldiretti, che si era schierata mentre gli agricoltori hanno votato no. Diciamolo agli industriali, la cui categoria si era schierata, mentre gli industriali veri, quelli che lavorano, quelli che hanno i calli sulle mani, invece dicevano di no. Mica gli amici del palazzo, amici degli amici degli amici. Agli amici degli amici degli amici hanno detto no. Gli italiani hanno detto no e quindi noi diciamo no a questa ennesima fiducia. Diciamo no alle marchette al signor De Luca e ai suoi amici contenute in questo disegno

Se lo ricorderanno gli italiani, quelli che vanno a votare, quando torneremo al voto, il più presto possibile. Renzi vuole andare al voto? Lo sfidiamo. Si ricorderanno, gli amici di Taranto, di quei 50 milioni che gli avete fottuto

e non basterà, cari colleghi della maggioranza (ditelo al presidente Renzi, che neanche ha avuto il coraggio di venire in quest'Aula almeno per l'ultima fiducia), fiducia), mettere un Governo, da chiunque sarà costituito, per poi trovarci il Presidente del Consiglio che si rifà una verginità, perché gli errori fatti in mille giorni di niente gli italiani se li ricorderanno e noi saremo il megafono che ricorderà loro di questi mille giorni di assoluto niente. Avete promesso una riforma al mese e non siete riusciti a mantenere la promessa.

Ci aveva presi in giro, il signore di Firenze, dicendo, se ve lo ricordate (nel 2014, quando avevamo iniziato a trattare le riforme costituzionali), che noi eravamo i capponi:

che quell'accozzaglia, come ci ha chiamati lui, ha tirato il collo al cappone. A casa, signori! A casa!

davanti quanto scrisse il «Sole 24 Ore»: «Secondo alcuni analisti tecnici la discesa della moneta unica europea a quota 1,05 potrebbe aprire ad un ribasso fino all'1,025 e da lì verso la parità nei confronti del biglietto verde». Mai una previsione fu così intempestiva. Quel movimento durò lo spazio di poche ore. Già all'indomani l'euro aveva ripreso il suo valore originario, iniziando una corsa al rialzo che ancora oggi non è terminata, fino a rivalutarsi del 2,5 Identico il movimento degli *spread* sui titoli italiani: rimasti sostanzialmente stabili, del tutto in linea con quanto avveniva negli altri Paesi dell'Eurozona. Lo stesso differenziale con i *bono* spagnoli - considerati il parametro di riferimento più indicativo - è rimasto più o meno fisso: intorno ai 50 punti base. Le cassandre del disastro annunciato sono state servite. Nessuna riedizione, quindi, della crisi del 2011. Nessun *Diktat* da parte della BCE di Trichet. Un baratro che potrebbe riaprirsi se sbagliassimo le nostre mosse, alimentando comportamenti irresponsabili, e scambiassimo la normale dialettica democratica, che si è sostanziata in un *referendum*,

*business as usual*, come dicono i britannici, ossia: «Niente di nuovo sul fronte occidentale», il bel libro di Erich Maria Remarque, prima che le milizie naziste lo mandassero al rogo. al rogo. In Italia c'è un'atmosfera cupa, la drammatizzazione di una situazione indubbiamente complessa, ma che non è certo il preludio di una catastrofe imminente. Un contrasto così evidente deve far riflettere, per evitare che ad errori si aggiungano altri errori, determinando una spirale - questa volta sì - senza controllo. Occorre quindi non cedere alle crisi di nervi, ma guardare con freddezza alla situazione che si è creata, andando oltre il ristretto perimetro del nostro operare, per misurarsi con i problemi di un Paese che ha dato dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, di una grande maturità democratica. Una partecipazione così alta non era né prevista né scontata. Come non lo fu quella del *referendum* sulla scala mobile, anche quella volta voluto - la storia che si ripete - dal Partito Un *referendum* che nuovamente ha dato voce al Paese più profondo, facendo emergere le ansie, il disagio, le incertezze del nostro popolo, ma anche la voglia di un nuovo protagonismo, la sua fiducia negli strumenti della democrazia, un capitale che non possiamo disperdere nei riti di una politica che sembra puntare solo ed esclusivamente

dato e chi ha avuto ha avuto. Tanto più che, come ho cercato prima di dimostrare, non c'è alcun Annibale alle porte e quindi abbiamo il tempo indispensabile per evitare il comportamento della gatta che, come ricorda il proverbio, acceca i propri figli. Naturalmente, questo non significa voler allungare il brodo, significa solo avere il tempo indispensabile per completare l'*iter* di un processo, la cui ingiustificata interruzione rischia di far più male che bene. E che l'interruzione sia ingiustificata è dimostrata dimostrata dallo stato delle cose: il presidente Renzi non ha ancora formalizzato le sue dimissioni e permettetemi solo di ricordare il comunicato del presidente Mattarella: «Vi sono di fronte a noi impegni e scadenze di cui le istituzioni dovranno assicurare in ogni caso il rispetto, garantendo risposte all'altezza dei problemi del momento». Impegni e scadenze. I due termini della questione non sono contrapposti, ma formano un *continuum* logico in cui l'aspetto qualitativo (ossia gli impegni) è ulteriormente rafforzato dall'ulteriore sottolineatura: «risposte all'altezza dei problemi del momento». Si rispetta questa indicazione, chiudendo in fretta e furia il *dossier* della manovra, per poi fuggire non si sa dove, pur avendo piena contezza della sua insufficienza e provvisorietà? Sarebbe il regalo più grande ai teorici dell'antipolitica. Lisciar loro il pelo: ecco i senatori che scappano di fronte alle loro responsabilità. Aver garantito con il voto del *referendum* l'esistenza del Senato della Repubblica, eletto su basi universali, è stato allora un errore? Dobbiamo evitare di fare questo regalo a chi non lo merita e dobbiamo dimostrare, al contrario, che i senatori della Repubblica si assumono pienamente le proprie responsabilità, anche se tutto ciò può alimentare, nell'immediato, qualche incomprensione

con passione e dedizione, anche se gli sforzi profusi si sono dimostrati insufficienti. Non è stato un lavoro inutile e lo vedremo nei prossimi mesi, quando la polvere delle polemiche e dei pretesti si sarà sedimentata. Con la stessa franchezza, tuttavia, non possiamo non vedere la crisi del partito di maggioranza relativa. Si deve ai suoi contrasti interni l'esito di questa legislatura e alla scarsa lungimiranza di chi ha maneggiato strumenti delicati come le primarie al di fuori del contesto istituzionale (la scelta del *leader* in prossimità di elezioni politiche) in cui tale meccanismo può e deve essere utilizzato. Da allora, infatti, il contrasto è stato permanente. Noi riteniamo che sia giunto il momento che il Partito Democratico risolva le sue contraddizioni, ma lo faccia senza travolgere le istituzioni, che devono rimanere il presidio più alto della volontà e delle libertà del popolo. Confidiamo in questo nella saggezza

Noi oggi dovevamo risolvere il problema dei 22.000 precari siciliani di enti e amministrazioni; dovevamo farlo nel corso del passaggio al Senato, perché la Camera non ne ha avuto il tempo. Ci auguriamo che lo faccia il prossimo Governo. A lui, cioè al Presidente della Repubblica, ci rimettiamo per le decisioni future. Non sarà un compito il tema più immediato e delicato, quello di una legge elettorale che non può essere affetta da strabismo: Camera e Senato, pur con le necessarie differenze, devono rispondere ad un identico schema concettuale e risolvere contestualmente il problema della governabilità e della rappresentanza. Per fortuna, come dicevo all'inizio, i mercati internazionali hanno mostrato una saggezza maggiore di tanti commentatori, la cui autorevolezza è stata messa in discussione. Sarebbe quindi paradossale che le fibrillazioni di un ceto politico totalmente immerso nella coltivazione del proprio orticello possano trasformare quella relativa calma in una tempesta tropicale. Da parte nostra ci facciamo carico di tutte queste contraddizioni. Questa legge di bilancio non ci piace e la sua incompiutezza è evidente: le delicate questioni lasciate in sospeso non potranno trovare le necessarie soluzioni. Ma non per questo faremo mancare il nostro voto, - sia ben chiaro - daremo solo alla luce della complessa situazione che si è andata delineando, nella speranza che questo nostro atteggiamento possa in qualche modo aiutare il presidente Mattarella nei compiti difficili che lo attendono, che sono compiti costituzionali che ci vengono dalla sovranità popolare, come

nel prenderne atto, con lo stesso senso di responsabilità che in queste ore guida l'operato delle nostre istituzioni, a partire dal Capo dello Stato e dal Presidente del Consiglio che ha congelato le proprie dimissioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale con quanto hanno fatto i nostri colleghi a Montecitorio. Sia ben chiaro, però, che voteremo la fiducia solo alla luce della complessa situazione che si è andata delineando, nella speranza che questo nostro atteggiamento possa essere d'aiuto al presidente Mattarella nell'applicare compito che la Costituzione gli assegna e che è stato riconfermato con forza dal popolo sovrano.

per evitare, ancora una volta, di affrontare le questioni vere del Paese. Ci è stato detto che bisognava fare di corsa, che non si poteva assolutamente modificare nulla, perché immediatamente dopo Renzi si doveva dimettere, che bisognava evitare l'esercizio provvisorio. Oggi scopriamo che le sue dimissioni sono rinviate probabilmente a venerdì,

con il modo in cui Renzi è arrivato a diventare Presidente del Consiglio? Forse ha paura di un'altra congiura di Palazzo che può sostituirlo con un altro magari non gradito? Certo, gli interrogativi sono tanti.

Il Presidente del Consiglio *smart*, che riceve più dell'80 per cento di «no» da parte dei giovani: questa dovrebbe essere la certificazione del fallimento del suo tentativo di scassare la nostra Costituzione, ma anche del fallimento di tutta la sua politica economica e delle politiche che ha messo in atto in questi tre anni, che hanno consegnato un Paese

ha permesso che le persone fossero umiliate. L'altro giorno sono stata colpita dal racconto di una ragazza che lavora da molti anni a un ristorante in questi ultimi due anni, proprio dopo l'approvazione del *jobs act*, non solo lavora con stipendi molto bassi (e magari si sente anche fortunata, perché almeno ha uno straccio di lavoro), ma,

Questo è il bilancio degli ultimi tre anni. I cittadini l'hanno fatto e sono stati molto più saggi dei giornali, delle televisioni e di tutti gli *opinion maker*. Hanno capito che dovevano dare un segnale forte e hanno respinto non solo quella riforma, ma queste ma queste scelte. Gli insegnanti: anch'essi umiliati con quella buona scuola. E non si è voluto sentire nessuno, si è umiliato anche questo Parlamento. Non si è mai voluto fare un ragionamento serio, accogliere proposte o discuterne. Anche oggi alla Camera si assumono degli impegni. Voglio citare qui la vicenda dei 50 milioni per i bambini dell'ILVA. Il "fu" Presidente del Consiglio ha persino sollevato polemiche, dicendo che avrebbero fatto la manifestazione il sabato, perché volevano strumentalizzarla ai fini del *referendum*. Si erano impegnati a stanziare i milioni dopo che lui aveva scelto di dare le risorse, 600 milioni, a De Luca, perché gli doveva portare i voti,

in cui bisognava annientare tutti, i corpi intermedi e la concertazione. Poi all'improvviso, qualche ora prima del *referendum*, riscopre che è importante la concertazione. Si accorge che da sette anni il pubblico impiego non ha il contratto rinnovato e quindi firma un preaccordo. Anche qui si impegna e anche questo doveva affrontare la manovra al Senato.

almeno provare a rimediare a tutta una manovra di bilancio che era stata pensata con trucchi. Pensiamo a tutte le vicende dei conti e dei saldi, a tutti i trucchi e trucchetti e alla propaganda elettorale per cui era stata confezionata. I cittadini italiani, soprattutto i giovani, gli hanno detto no, perché - torno a

Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie condivide e sostiene la decisione del Governo di porre questa fiducia un po' atipica, detta anche tecnica, per l'approvazione del disegno di legge di bilancio. di una scelta di responsabilità, in considerazione della grave crisi politica e di governo imposta dall'esito purtroppo negativo del *referendum* costituzionale. Anche noi, senatori del Gruppo Per le Autonomie, avremmo preferito l'esame del disegno di legge di bilancio anche da parte del Senato, ma non si può non tener conto e riconoscere le priorità politiche e istituzionali che richiedono un'urgente conclusione dell'*iter* parlamentare della manovra di bilancio per il 2017, anche per salvaguardare i saldi di finanza pubblica.

Ricordo che tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione hanno chiesto il *referendum* affinché si esprimessero i cittadini. la riforma è stata apprezzata: in provincia di Bolzano quasi due terzi degli elettori si sono espressi a favore del sì, ma purtroppo è andata diversamente a livello nazionale e quindi ora si aprirà

come ha fatto nel corso della sua breve esperienza di Governo: lo apprezziamo e ne condividiamo sia le ragioni, sia la scelta ultima di rassegnare le dimissioni. il Governo Renzi ha operato bene, ha varato importanti riforme come il *jobs act*, la riduzione delle imposte e l'alleggerimento del peso fiscale sulle imprese. Penso che avrebbe dovuto andare avanti, ma purtroppo non è andata così. Come rappresentanti delle Autonomie speciali abbiamo profondamente apprezzato la sensibilità che il Governo Renzi ha costantemente avuto nei nostri confronti. C'è stato un percorso di grande collaborazione e i progressi graduali, ma costanti, che il Governo Renzi ha compiuto insieme a noi, ci hanno consentito di superare problemi

ma presenta anche le basi per una rinnovata fase di sviluppo delle nostre Autonomie, che la riforma costituzionale avrebbe rafforzato,

Ora si impongono valutazioni e considerazioni certamente difficili in ordine alla situazione politica e di Governo derivante dall'esito referendario. Come Gruppo per le Autonomie siamo pronti a sostenere un Governo di responsabilità istituzionale e che sia in grado di garantire un sistema omogeneo di voto, per la Camera dei deputati e per il Senato, anche in base alle decisioni che assumerà la Corte costituzionale in merito all'Italicum. Siamo nettamente contrari ad un salto nel buio, perché pensiamo che gli italiani hanno bisogno di tutto, ma certamente non

In questo senso speriamo che le scelte del presidente Mattarella andranno in questa direzione. Concordiamo sul fatto che, nell'attuale situazione, le necessarie scelte di responsabilità chiamino in causa tutte le forze politiche, non solo quelle che

dopo i cittadini possano almeno andare a votare con una certa tranquillità. Poi vinca chi deve vincere, però almeno sulle regole, come

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando sono entrato per la prima volta in questo Parlamento, a marzo 2013, immaginavo che economia e lavoro fossero le priorità dell'azione di Governo. Mi sono dovuto ricredere e oggi sono francamente allibito dal fatto che sembra che non sia successo nulla. Infatti, peraltro, nessuna delle tragedie che sarebbero dovute accadere a seguito della vittoria del no alla scriteriata riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi si è verificata, è accaduta o si è avverata. È accaduto, invece, che il popolo italiano ha sonoramente schiaffeggiato questo Governo, bloccandone il poco credibile operato. Cosa è successo nella sostanza? Si è smontato il credo renziano della narrazione, signor Presidente. Gli italiani si sono incaricati di dire a Renzi quello che, purtroppo inascoltati, noi ripetiamo da tempo e cioè che la realtà nella quale il Paese vive è altra cosa rispetto alla narrazione renziana. Per un attimo era parso che il colpo fosse andato a segno, quando il Presidente del Consiglio aveva annunciato le sue dimissioni al Presidente della Repubblica. Ma come sempre nelle strategie e nelle logiche di Matteo Renzi c'è sempre un anodino retro pensiero. Buono a nulla ma capace di tutto, avrebbe detto Leo Longanesi, e infatti sta tutto nella sua diabolica logica l'*iter* che questo disegno di legge di bilancio sta attraversando. Accade, cioè, che un Governo dimissionario venga nell'Aula del Senato, un'Assemblea oggi ancora più forte nella sua autorevolezza a seguito del recente voto degli italiani, e venga a chiedere la fiducia. Nella sostanza, Renzi e il suo Governo oltraggiano, ancora una volta, le istituzioni del nostro Paese, la volontà degli italiani e - mi consenta, mi permetta - la nostra intelligenza. Noi siamo qui a discutere della più importante legge che ci tocca licenziare ogni anno in questo scenario, signor Presidente, desolante: un'Aula semideserta e, quel che è peggio, tale soprattutto nei banchi della maggioranza perché i parlamentari di maggioranza sono impegnati a capire quale sarà, a seguito delle dimissioni di questo Governo, il loro personale futuro. Confermano, cioè, che delle sorti del Paese a loro importa poco o nulla, come ha mirabilmente rappresentato il Ministro dell'interno quando, dimenticando ruolo e funzione, ha anche annunciato il voto di febbraio, dimenticandosi peraltro che c'è anche un Presidente della Repubblica, ma forse qualcuno non gli ha ancora comunicato che la riforma costituzionale non è passata. A loro importa sostanzialmente della direzione del Partito Democratico, direzione nella quale arrivare con il bottino rappresentato dalla legge di bilancio.

non so se posso usare il termine perché mi è stato più volte rimproverato - di marchette elettorali. Eccola smascherata la narrazione renziana. Questo provvedimento è la somma di tutte le sue bugie, e mi auguro sia l'ultima. - scusate, votano - leggi di bilancio totalmente a debito, in modo totalmente irresponsabile, senza che alcuno gridi allo scandalo, sino ad arrivare a quest'ultimo disegno di legge di bilancio pieno di spese senza copertura, che spende altra flessibilità: quello del quale, a ragione, si lamenta l'Unione europea. E perché si lamenta l'Unione europea? Perché nessuna delle previsioni di questo Governo in questi tre anni si è avverata. La situazione economica è peggiorata di anno in anno e il risultato, che nessun organo di stampa e di comunicazione si azzarda a comunicare, è che il Governo Renzi ha aumentato il debito pubblico di centocinquanta miliardi e ha azzerato l'avanzo primario del nostro Paese. Ecco nella narrazione renziana cosa lascia in eredità ai nostri figli questo Governo. Dovremo faticare per evitare che scattino le clausole di salvaguardia e, al contempo, dovremo raccogliere le macerie istituzionali, dovremo sanare gli sfregi ai Regolamenti parlamentari, dovremo, in buona sostanza, recuperare ragione all'arrogante e scriteriato abuso al quale sono state sottoposte le nostre istituzioni. Per far questo, signor Presidente, il nostro Gruppo inizierà negando la fiducia a questa ultima (ci auguriamo sia l'ultima) farsa parlamentare.

dicevamo prima, la fretta era importante. Noi, come Gruppo di opposizione, avevamo predisposto, nonostante la campagna referendaria e sapendo che i tempi erano ristretti, un migliaio di emendamenti.

concesso. Rattrista anche vedere che questo Governo, invece di perseguire gli interessi dei cittadini, ha perseguito gli interessi di società finanziarie, di strutture internazionali.

Spero davvero sia finita questa narrazione - come si diceva - perché in queste settimane ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori: dal fatto che con questa "schiforma"

vedo che più di 100.000 ragazzi all'anno lasciano questo Paese per andare all'estero. Questo secondo me è il dato più importante. In un dato solo si riassume

davvero accettato di buon grado di vedere un minimo di umiltà, e invece ho notato ancora l'arroganza di queste persone: l'esempio del ministro Boschi che viene qui a chiedere la fiducia, proprio lei che è stata l'artefice di una "schiforma" che gli italiani hanno bocciato in maniera così pesante. Mi sarei aspettato anche un passo indietro di qualcun altro come il vero artefice di questa situazione, il presidente Napolitano. Napolitano. Mi sarei aspettato una sua dichiarazione, quantomeno un *mea culpa*: spero ne prenda atto e che quantomeno abbia la dignità di non presentarsi in questo Senato fortemente legittimato dai cittadini italiani.

proprio per il fatto che non avete voluto capire che gli italiani hanno bisogno, che gli italiani ci stanno chiedendo aiuto, che si trovano in difficoltà. I numeri sono già stati detti in questa sede e non li ripeto, ma non capire fino in fondo questo, per un professionista della sanità, per uno che si occupa dei bisogni delle persone, veramente mi ferisce, non solo come politico, non solo come professionista, ma soprattutto come cittadino. È veramente indecente che accettiate questo tipo di situazione, per un Presidente del Consiglio ci ha fregato per tre anni e che veramente non lo merita. apre una nuova finestra"). Vorrei ricordare che tutti i componenti di questa Assemblea sono egualmente legittimati a pieno titolo a prendere parte alle sedute. [ROMANI

queste sono le parole con cui Matteo Renzi presentava il suo Governo in quest'Aula il 24 febbraio 2014. Oggi, dopo 61 voti di fiducia nelle due Assemblee, siamo arrivati, grazie alla volontà degli italiani, al capitolo finale: finale per il Governo Renzi, non certamente per il Senato. Voglio soffermarmi brevemente su questo disegno di legge di bilancio su cui avete posto la questione di fiducia tecnica, visto che alcuni colleghi non hanno nemmeno fatto la dichiarazione di voto, malgrado siate stati sfiduciati dal Paese e il vostro sia un Governo presumo dimissionario. Poi le dimissioni non si sa se saranno secondo le notizie delle ultime ore, sembra che verranno date venerdì. Vorremmo sapere nel frattempo che cosa dovrebbe accadere. Nonostante questo, avete deciso ancora una volta di non affrontare serenamente il giudizio della Commissione bilancio prima e dell'Assemblea poi. Il perché è abbastanza evidente: avete composto un disegno di legge di bilancio quasi esclusivamente elettorale, impegnati a cercare di raggranellare i consensi più disparati in vista del *referendum* piuttosto che per fare il bene dell'Italia. Oltre alla scontata eliminazione della clausola di salvaguardia sull'IVA per 15 miliardi, non si riesce a vedere alcuna strategia, alcuna priorità, alcun ragionamento sul sistema Paese. Altri prima di me hanno già smontato nel merito questo pessimo disegno di legge di bilancio ed io voglio aggiungere solo una cosa. La stessa maggioranza sa benissimo che occorreva rimetterci le mani: solo ieri, il vice ministro Morando citava le norme sull'ecobonus e sulle ristrutturazioni, i problemi legati all'ILVA, agli sgravi per i terremotati, alla ripartizione del Fondo unico per gli enti locali come argomenti che avrebbero avuto bisogno di una soluzione in questo passaggio al Senato e che invece si risolverà con l'ennesimo voto di fiducia. Il nostro giudizio su questa legge di bilancio non può quindi che essere di netto dissenso, per il metodo e ancora di più per i contenuti. Ma mi preme Ma mi preme anche fare qualche considerazione sulla fine dell'esperienza di questo Governo. Nelle prossime ore, auspicabilmente, il Primo Ministro consegnerà nelle mani del presidente Mattarella le sue dimissioni (riteniamo irrevocabili). Lo farà perché il giudizio che gli italiani hanno dato sugli oltre mille giorni del suo Governo è chiaro e inappellabile: per cento dei nostri concittadini, con una partecipazione del 70 per cento, ha detto un forte no ad una riforma pasticciata, che ha via via perso per strada le ragioni di condivisione e di discussione comune; un progetto di revisione che doveva essere condiviso e che è riuscito solo a spaccare il Paese. Una riforma imposta dal Governo, quando un Governo dovrebbe astenersi anche solo dal partecipare, come ricordava Piero Calamandrei: «Nel campo del potere costituente il Governo non può avere alcuna iniziativa, neanche preparatoria»; e ancora: «Quando l'Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del Governo dovranno essere vuoti». Il popolo italiano ha detto no anche al tentativo, attuato con il combinato di Italicum, dell'eliminazione delle Province (una finta eliminazione, che ha eliminato il voto popolare e creato una marea di nuovi problemi di competenze), della nomina governativa della dirigenza RAI e dell'impianto complessivo della riforma, con cui si è cercato di imporre una forte e pericolosa diminuzione degli spazi di democrazia nel nostro Paese. Ma io credo che il popolo italiano abbia detto «no» anche e soprattutto ad un Governo ricco di *slide* e povero di idee, che non ha saputo far ripartire il nostro Paese e non è stato in grado di dare speranza per il futuro dei nostri concittadini. Un Governo che ha fallito in ognuna delle grandi riforme che ha voluto affrontare. Ad esempio, il *jobs act*, le cui buone intenzioni iniziali sono state subito annullate dalle resistenze interne al Partito Democratico, rendendolo un provvedimento debole e contradditorio, che ha portato risultati discutibili in termine di nuova occupazione, comunque inferiori alla media europea e drogati dagli incentivi temporanei. Poi la buona scuola, che di buono ha ben poco, e che si è risolta in una assunzione di massa, senza alcun progetto e senza riuscire a cambiare la qualità della scuola italiana. Ancora, la riforma della pubblica amministrazione, miseramente arenata sugli errori evidenziati dalla Consulta, e la riforma della Giustizia, che stiamo ancora aspettando. Un Governo che non ha avuto né il coraggio né la capacità di affrontare il problema del debito pubblico italiano, nascondendosi dietro la riduzione del costo del servizio del debito, che è stato generato, non certo per merito del Governo, dalla diminuzione dei tassi. Un Governo che ha dimostrato pochissima capacità in politica estera, indeciso su tutto, incapace di affrontare alla radice il problema dell'immigrazione e della tratta degli esseri umani, che non ha saputo incidere sulle aree di crisi, neanche quelle che sono di riconosciuta competenza italiana come la Libia. che ha passivamente seguito la politica suicida europea della contrapposizione con la Russia, che infine ha dato un inopportuno e plateale appoggio alla candidata Clinton, rischiando di mettere in discussione i nostri consolidati rapporti con il più importante degli alleati. che ha avuto con l'Unione europea un rapporto debole e perdente, nascosto dietro i muscoli della violenza verbale. Un Governo, infine, che ha inchiodato l'intero Paese su una interminabile campagna referendaria, rispetto alla quale tutti i reali problemi sono stati messi in secondo piano: immigrazione, sicurezza, tasse, e perfino terremoto. La fotografia che l'ultimo rapporto CENSIS dà di quest'Italia è impietosa: un Paese rinchiuso su sé stesso, con 15 milioni di persone povere o sulla soglia della povertà, disunito, disgregato e disperato. Guardate i risultati di questo *referendum*, la cui campagna allarmista è stata centrata sui pericoli dello sfascio, dei mercati, della tragedia che sarebbe seguita alla vittoria del no.

Non ci poteva essere altra risposta ad una politica che per il Sud non ha fatto niente, se non interventi *spot* e di emergenza. Dove è finito il grande piano strategico per il meridione d'Italia che Renzi aveva più volte promesso? E veramente la questione dei giovani, fondamentale per il futuro del nostro Paese, poteva essere affrontata solo con una *card* da 500, euro da spendere per andare al cinema o a teatro? Il dramma della disoccupazione giovanile, soprattutto al Sud, gli ascensori sociali che non funzionano più, intere generazioni che vivono nella precarietà, che sanno che il loro futuro sarà peggiore di quello dei loro padri.

Con quest'ultimo voto di fiducia tecnica e con le dimissioni del Presidente del Consiglio si apre una nuova pagina politica. Questo Governo ha operato fin dall'inizio in maniera divisiva, rifiutando ogni mediazione con i corpi sociali ed ogni possibilità di confronto, alienandosi le simpatie di intere categorie (insegnanti, giovani, sindacati, pensionati); non ha saputo dare risposte alla povertà ed alla disperazione sociale, non ha saputo affrontare il nodo delle banche e dei correntisti che hanno perso tutti o quasi tutti i loro risparmi, si è scordato del Sud e delle piccole imprese, spina dorsale dell'impianto produttivo del nostro Paese. Questo Governo è rimasto isolato, con a fianco solo alcuni poteri forti, o presunti tali, che forse così forti non sono più: i grandi giornali, la Confindustria, la Coldiretti, le grandi banche e poco altro. Guardate la reazione dei mercati alla notizia delle sue dimissioni e capirete quanto poco sia in sintonia con il resto del Paese. E oggi la maggioranza pretenderebbe che qualcuno venisse in suo soccorso,

Del resto, per noi il percorso è chiaro e obbligatorio. È necessario dare all'Italia il prima possibile una legge elettorale ragionevole, che sappia garantire la governabilità ma anche una reale rappresentazione del Paese. Subito dopo si potrà finalmente ridare la parola agli italiani, dopo tre Governi che non hanno avuto un'investitura elettorale. *(Applausi dal Gruppo perché sappiamo che solo una proposta politica seria e responsabile come quella di Forza Italia e di tutto il centrodestra - lo ribadisco: di tutto il centrodestra - basata sulle reali necessità dei cittadini e delle forze produttive, sulla capacità di unire e non di dividere, sia in grado di rilanciare il Paese e sia l'unica risposta credibile alla crisi globale ed alla debolezza della rappresentanza politica.

voterà la fiducia al Governo affinché si possa approvare il disegno di legge di bilancio che definisce il quadro economico per il 2017 e poi anche per gli anni successivi. È un atto di responsabilità e di tutela per il Paese perché occorre ricordare che, senza l'approvazione della legge di bilancio, da gennaio 2017 entrerebbe in vigore l'esercizio provvisorio soprattutto dal 1° gennaio, scatterebbero imposte per oltre 15 miliardi su IVA e accise che avrebbero gravato ulteriormente la vita già difficile dei nostri concittadini. È un atto di responsabilità verso il Paese che vuol contribuire a rendere meno ostica la soluzione della crisi politica che si è aperta con le dimissioni del Governo e che da domani potrà essere affrontata dal Capo dello Stato e dalle diverse forze politiche senza la pesante ipoteca che sarebbe stata rappresentata dall'incertezza del quadro economico. In questo senso l'approvazione del disegno di legge di bilancio dà un quadro di riferimento anche ai rapporti con l'Unione europea che, diversamente, sarebbero sostanzialmente lasciati ad un'unica decisione da parte delle autorità dell'Unione europea. In tale ottica, senza entrare nel merito dei singoli temi e sforzandoci di non ricadere nel facile esercizio - che abbiamo sentito anche stamane - della polemica interessata, ci sono in questa legge di bilancio a suggello di una legislatura di riforme provvedimenti di natura strutturale che vanno nella giusta direzione di irrobustire il percorso difficile per la ripresa dell'economia, del lavoro e delle politiche di contrasto alla povertà, che hanno segnato già dagli scorsi anni le scelte del Governo in questa legislatura e sono state necessarie perché - forse adesso non lo si ricorda più - questa legislatura è iniziata con una recessione molto grave, con la disoccupazione a livelli altissimi, con la finanza pubblica in grande difficoltà. Ho parlato di interventi strutturali. Si prosegue con questa legge di bilancio nel cammino di riduzione della pressione fiscale in capo alle diverse realtà del mondo produttivo (le piccole imprese, le imprese individuali, le società, le *start up*, le partite IVA, il mondo agricolo) per diminuire, dopo gli interventi realizzati negli scorsi anni, la tassazione sul lavoro e sulle famiglie. Si rafforza, sempre in via strutturale il sostegno agli investimenti privati, vero punto ancora irrisolto nel nostro Paese, con la riproposizione del superammortamento (con un allargamento anche agli investimenti digitali), con il credito d'imposta per il Sud e per la ricerca, con l'ampliamento del fondo di garanzia per i crediti. Si prosegue la riduzione degli oneri contributivi sul lavoro soprattutto per i giovani e per il Sud, in attesa, nel 2018, di un intervento strutturale in tutto il settore del lavoro. Si caratterizzano gli investimenti pubblici con la predisposizione di fondi pluriennali dedicati sia alle infrastrutture sia alla sicurezza sismica e idrogeologica sia alla gestione delle emergenze, in modo tale che questi investimenti pubblici siano soggetti ad un percorso crescente di impatto con le diverse esigenze di messa in sicurezza, di innovazione, di rafforzamento di tutte le infrastrutture fondamentali del nostro Paese. Si favorisce con gli ecobonus il risparmio energetico e il rinnovamento del patrimonio abitativo delle famiglie anche con forti innovazioni, come per quanto quindi un intervento che, ripeto, completa un percorso di riforme che non ha avuto certamente l'esito catastrofico qui enunciato, ma importanti risultati e soprattutto ha permesso di conseguire un segno positivo per la nostra economia, un segno positivo per quanto riguarda il lavoro. Vi è un segno positivo anche per quanto riguarda il capitolo delle politiche sociali, dove possiamo registrare interventi che aiutano, da un lato, le pensioni più basse e aprono, dall'altro, con la necessaria prudenza, una flessibilità pensionistica

in tempi certi - nessuno lo ha detto, perché non dirlo? - il superamento del Patto di stabilità per gli enti locali e le Regioni, che potranno ora disporre, anche con questa legge di bilancio, di un fondo dedicato da ripartire tra Province, enti locali e Regioni,

sul favorire le nascite, sul contrasto alla povertà, che sono stati avviati e che hanno bisogno ora di essere continuati anche nei prossimi anni. di legge di bilancio completa sul piano economico un percorso che è partito da un Paese in grave recessione, il quale ha iniziato invece dal 2013, nel 2014, nel 2015 e nel 2016, a riprendere a camminare e a dare segnali importanti e positivi, che vanno consolidati. il Paese ha necessità di uscire dalla crisi politica. Lo deve fare ritrovando innanzitutto una capacità di collaborazione istituzionale, per definire rapidamente regole certe, per avviare rapidamente una nuova fase nella quale le forze politiche, sulla base di un consenso elettorale dei cittadini, possano riprendere il testimone della guida politica, per proseguire, completare e migliorare quanto fatto in questi quattro anni. Abbiamo la piena convinzione di consegnare al Paese, con la legge di bilancio, un quadro di provvedimenti necessari e utili a proseguire questo cammino e a farlo nell'interesse di tutti i nostri cittadini, per portare il Paese verso risultati ancora migliori, che giustamente dobbiamo tutti quanti contribuire a costruire. Per questi motivi il Gruppo del Partito Democratico vota con convinzione la fiducia al Governo.

votazione nominale con appello dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2611, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Latorre. SCOMA,

una nuova finestra"). Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2611, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

La Presidenza dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 138, comma 6, del Regolamento gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.10, in quanto recano disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente. Tali emendamenti sono in ogni caso preclusi per effetto dell'approvazione dell'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, con l'annessa tabella.